Faccio riferimento al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza. La eterogeneità è motivo di preoccupazione per molti di noi. L'articolo 10 del Patto della salute prevedeva un aggiornamento del monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza; ci domandiamo a che punto siamo e quali sono i nuovi criteri. criteri. Con riguardo alla continuità e alla qualità dell'assistenza garantita alle persone che soffrono di patologie croniche, c'è il problema di garantire la personalizzazione soprattutto dei presidi e dei prodotti monouso.

è possibile) qualche elemento che faccia riferimento esplicitamente - forse più di quanto non sia già attualmente - alla qualità dei presidi e non soltanto al costo, come previsto dall'articolo 67 della direttiva europea. La preoccupazione riguarda poi la sicurezza in presenza di tanti rischi che abbiamo soprattutto sui sistemi informativi e ICT, anche per le infrastrutture critiche sanitarie. Vorremmo sapere, riguardo alle strutture sanitarie che sono considerate dall'Unione europea infrastrutture critiche,

vengo all'interrogazione relativa ai livelli essenziali di assistenza. Signora Ministra, lei, nelle comunicazioni che ha reso alla Commissione sanità nel giugno 2013 sulle linee programmatiche del suo Dicastero, annunciava essere *in itinere* la revisione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e rilevava come risulti prioritario definire un nuovo patto per la salute quale piano regolatore della sanità. A tre anni di distanza quella revisione rimane tutt'ora non attuata, come rimane una profonda sperequazione a danno dei cittadini tra i livelli essenziali È un problema che rimane irrisolto, e aggiungo - siccome voglio essere onesto - da oltre un decennio, la cui mancata risoluzione non può essere imputata solamente a lei, che tra l'altro ha annunciato a fine febbraio un'imminente emanazione dei nuovi LEA. Oltre alla richiesta di fornire notizie sullo stato dei fatti relativo alla revisione dei livelli essenziali di assistenza, le pongo due questioni, signora Ministra. Può dare maggiori indicazioni su come monitorare la spesa farmacologica, affinché nelle terapie possa essere riservato eguale accesso a tutti i cittadini, in modo da conseguire maggiori risparmi e, al contempo, sostenere l'industria farmaceutica nazionale? Come seconda domanda vorrei sapere quale sia la posizione del suo Dicastero sul tema rilevante delle malattie rare,

Signor Ministro, mi collego all'intervento del senatore Zuffada proprio per ricordarle che questo ramo del Parlamento ha approvato, in sede deliberante, il disegno di legge Atto Senato 998, che disciplina l'inserimento nei degli *screening* neonatali. Questo provvedimento, approvato a larga maggioranza, anzi all'unanimità, da parte di tutte le forze politiche, è ora in discussione alla Camera. L'inserimento degli *screening* all'interno dei LEA è l'unica maniera per garantire che la diagnosi precoce risolutiva di patologie metaboliche possa essere applicata su tutto il territorio nazionale. Mi permetto di dirle che, in spregio a tutte le basilari norme di correttezza istituzionale, questo Ministero si vede oggi promotore di un decreto che è in netto contrasto con il il principio fondamentale del disegno di legge approvato al Senato. In particolar modo è in contrasto perché prevede un contenuto fortemente deteriore: tale *screening* non viene inserito nei LEA, non diventa obbligatorio e rimane in un'area di sperimentazione totalmente inutile, considerando che gli *screening* vengono fatti in Toscana già dal 2004 e che tutta la comunità scientifica ne riconosce la totale validità. Perché, allora, scavalcare l'organo deputato a legiferare proprio quando è arrivato a un passo dall'approvazione definitiva della legge? Perché introdurre uno *screening* parziale, inefficace e portatore delle medesime differenziazioni regionali che da anni attanagliano la sanità? Signor Ministro, vorrei parlare di vaccini, perché i dati del Ministero 2013-2014 ci dicono che le coperture sono

Aggrediamo anche la situazione delle Regioni perché purtroppo ci troviamo di fronte anche a diseguaglianze di copertura Regione per Regione. Personalmente, ritengo che vaccinare sia interesse superiore del fanciullo e che l'immunità di gregge contro le malattie prevedibili con i vaccini sia un bene pubblico che non possiamo escludere dai nostri piani sanitari. Signor secondo lei, deve prevalere la decisione dei genitori di non vaccinare rispetto al diritto di un bambino ad essere protetto mediante le vaccinazioni? Il diritto-dovere di ogni genitore ad allevare i propri figli giustifica le decisioni che pongono la comunità a rischio? luogo, il piano vaccinale del suo Ministero cosa prevede per una buona comunicazione, per un cambio di rotta culturale, per un maggiore coinvolgimento del personale sanitario? Infine, possiamo sfatare definitivamente e scientificamente che l'autismo non può e non deve essere considerato come effetto-conseguenza delle misure vaccinali? PRESIDENTE.

quando il Patto per la salute 2013-2015 ha sottratto alla sanità oltre 30 miliardi di euro, in un modo o in un altro i tagli si sono susseguiti in tutte le leggi di stabilità. Anche l'ultima, non è da meno: introduce una nuova tagliola sanitaria che porterà ad un'ulteriore riduzione delle prestazioni ai cittadini, attraverso i piani di rientro triennali per le aziende ospedaliere; inoltre di risparmiare riducendo ancora i prezzi unitari di acquisto. Pochi giorni addietro l'Associazione chirurghi ospedalieri italiani (ACOI) ha denunciato il livello qualitativamente basso dei bisturi ad uso del personale sanitario; denuncia cui si deve affiancare quella presentata nei mesi scorsi dalla Società italiana di chirurgia, che aveva segnalato l'impiego di guanti in lattice qualitativamente scadenti, o ancora la denuncia relativa ai misuratori di glicemia non funzionanti. Ma non sono solo i tagli per le forniture ad inficiare il corretto funzionamento del sistema sanitario; anche la mancanza di personale è un problema che si sta manifestando in tutta la sua portata. Infatti, per supplire alla grave carenza di personale (60.000 unità in meno rispetto al fabbisogno spesso si è reso necessario il ricorso a turni aggiuntivi in orario straordinario, tali da non consentire il recupero psicofisico, pregiudicando in tal modo i livelli di sicurezza sia del personale sia dei pazienti, e rischiando, tra l'altro, l'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Unione All'insufficienza del personale si deve necessariamente aggiungere anche quella delle strutture. I servizi territoriali sono di fatto inesistenti: non c'è nessuna struttura intermedia tra il medico di base e i nosocomi. I cittadini sono obbligati a rivolgersi agli ospedali dove la sistematica razionalizzazione dei reparti sta generando il caos: i posti letto vengono di anno in anno decurtati, creando una situazione tale che, in caso di necessità, i pazienti si trovano in reparti diversi da quelli di competenza, con assistenza, ovviamente diversa, quando non vengono collocati con una sistemazione di fortuna in altre stanze o corridoi, o addirittura nelle barelle quando non vi sono più letti disponibili. Queste condizioni indecorose costano la vita dei nostri cittadini, come nei casi - cito solo l'ultima settimana - della donna di Napoli, morta perché le sale operatorie erano occupate, o ancora quello del quarantunenne, sempre di Napoli, con un'emorragia alla testa è morto perché la TAC era rotta da giorni. La domanda è dunque: cosa si intende fare per ovviare a questa situazione in cui i nostri cittadini perdono la vita per via dei tagli sistematici che stanno riducendo all'osso il sistema sanitario? Fateci sapere se l'intento è quello di privatizzarlo, così smettiamo di prenderci in giro. UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Ministro, la sensibilità chimica multipla è una patologia controversa e complessa per l'inquadramento come entità ben

in assoluta difficoltà fino alla limitazione degli stessi contatti con i familiari, se non con particolari precauzioni e materiali protettivi. Per le sue condizioni, e per tutti i malati con sensibilità chimica multipla, è stata sottoscritta una petizione con circa 15.000 adesioni a sostegno: una partecipazione collettiva, corale, spontanea e, soprattutto, solidale. Le evidenze scientifiche, allo stato attuale, evidenziano un quadro contraddittorio, una condizione non ben definita e unica. Parimenti sono consapevole della necessità di non incorrere in facili speranze. Nel 2008 la seconda sezione del Consiglio superiore di sanità ha ritenuto che la indisponibilità di evidenze scientifiche non consentisse, Signor ministro Lorenzin, le chiedo di intervenire sulla questione che ho posto alla sua attenzione, anche interpellando il Consiglio superiore di sanità per rivalutare la sindrome da sensibilità chimica

ha un'origine di carattere economico: il fine ultimo è quello di alleggerire la spesa del sistema sanitario nazionale. Esso viene molto spesso infiorato come un approfondimento delle questioni scientifiche e mediche, ma così non è; non avviene per sua colpa, ma per il fatto che il Ministero della salute continua a soggiacere sotto l'imperio del Ministero dell'economia e delle finanze. Lei ha emanato questo decreto sull'appropriatezza dove sostanzialmente si è limitata, attraverso i tecnici, a restringere il novero delle prestazioni erogabili all'utenza. È stato fatto senza un *background* scientifico, senza descrivere l'evidenza scientifica e solamente per mettere più tempo tra gli intervalli delle prescrizioni di cui può usufruire il cittadino rispetto quelle che, in effetti, si aveva l'abitudine di prescrivere. Le faccio un esempio per mostrare con quanta pedestre modalità è stato fatto questo decreto.

La pubblicità del servizio non è la statalità della gestione. Lei ha un sistema sperequato: da una parte paga a tariffa, a prezzo prederminato e, dall'altra, paga a piè di lista.

Signor Presidente, i livelli essenziali di assistenza (LEA), vale a dire le prestazioni che il Servizio nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale, sono stati definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2001. I LEA sono organizzati in tre grandi aree: assistenza sanitaria, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. È molto importante ricordare che le prestazioni e i servizi inclusi nei LEA rappresentano il livello essenziale garantito a tutti i cittadini, ma le Regioni, come hanno fatto fino a oggi, potranno utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelli inclusi nei LEA. Il nuovo Patto per la salute 2014-2016 ha previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, in attuazione di principi di equità, innovazione e appropriatezza e nel rispetto degli equilibri programmati dalla finanza pubblica. Successivamente, la legge di stabilità 2015 ha ratificato in via normativa i contenuti del Patto per la salute. Con la legge di stabilità 2016 il Governo ha deciso di tagliare le risorse destinate al Fondo sanitario nazionale, che nell'anno dovrebbe attestarsi su 111 miliardi di euro, contro i 113 miliardi promessi inizialmente alle Regioni; di questi, 800 milioni di euro vengono vincolati per l'atteso aggiornamento dei LEA. le chiediamo se, essendo a conoscenza della situazione, non intenda intervenire reintegrando quanto tolto al comparto sanità, al fine di dare una piena e compiuta attuazione all'aggiornamento dei LEA, il cui rinnovamento appare indispensabile e urgente, senza togliere risorse indispensabili per il funzionamento dell'assistenza medica, soprattutto in quelle Regioni in cui il sistema sanitario è in equilibrio finanziario.

che i nostri cittadini ricevono presso il Servizio sanitario nazionale, non avveniva dal 2001, ossia da circa sedici anni. Le motivazioni per cui questo aggiornamento tardava ad arrivare sono molto semplici, in quanto non si riusciva a trovare un modello per garantire la copertura delle

Le griglie sono state riapprontate secondo un metodo di efficacia ed efficienza del sistema e tenendo conto anche di un meccanismo ormai acclarato

abbiamo dovuto attendere i dati delle Regioni, perché abbiamo dovuto fare un ulteriore monitoraggio volto a verificare quello che di questi LEA è stato già applicato

lungo *iter* di aggiornamento e di confronto, con i dati delle Regioni, è terminato; mancano ancora in realtà tre Regioni, ma noi possiamo dirci soddisfatti e siamo pronti a mandare il testo per il concerto al Ministero dell'economia e delle finanze. Quindi possiamo dire che l'*iter* si è di fatto concluso e credo che questa sia un'ottima notizia per i nostri cittadini. Ma ancora di più è un'ottima notizia il fatto che abbiamo finalmente reso

di come i dati sensibili vengono gestiti, trattati e mantenuti in sicurezza. Il dato è la vera forza economica dei nuovi sistemi dal punto di vista mondiale; su questo noi abbiamo dei protocolli, come Ministero della salute, con le autorità preposte al controllo e al monitoraggio dei sistemi informatici. Questo per noi è estremamente importante. È evidente che nel futuro tutti noi saremo impegnati, man mano che i dati diventeranno centrali nella gestione del nostro del nostro sistema, a fare in modo che i dati siano sicuri e siano soprattutto ben gestiti. Nelle altre domande che sono state poste da chi mi ha preceduto entra anche il tema della cronicità. La cronicità è una questione assolutamente di primo rilievo e fa parte non solo del piano di prevenzione, ma anche dei vari piani piani che stiamo predisponendo con il Ministero della salute su questo argomento. Nel nuovo Piano nazionale della cronicità abbiamo messo al centro proprio la presa in carico del paziente; da questo punto di vista, anche per quanto riguarda gli ausili e il nomenclatore, noi lavoriamo in modo tale che sia sia garantita la qualità della prestazione erogata al paziente cronico. Curare e trattare nel modo più appropriato il paziente cronico è ovviamente una sfida per i servizi sanitari nazionali moderni, in una società con un'alta presenza di persone della terza e della quarta età. Di fronte all'invecchiamento della popolazione, la sfida della cronicità è anche una sfida di sostenibilità.

Il mio precipuo interesse ed obiettivo, e quello di tutto il Governo, è mantenere il nostro Servizio sanitario nazionale come un modello universale e universalistico, che è la nostra grande differenza rispetto a quello che accade nella maggior parte dei Paesi del mondo. Quello che abbiamo in Italia, cioè accesso a cure e a prestazioni di massimo livello e di massima eccellenza in modo gratuito per a prescindere dalla propria carta d'identità e dalla propria carta di credito o dal fatto di avere o meno un'assicurazione privata, è una ricchezza sociale del nostro Paese. Questo tra l'altro lo facciamo spendendo pochissimo rispetto ai nostri altri vicini di casa: noi spendiamo il 6,5 per cento del prodotto interno lordo. Tutti ci chiedono: ma come fate? È ovvio che, per farlo, sono stati fatti grossi sacrifici in anni di crisi economica. Ma, a differenza di altri, durante la crisi economica noi non abbiamo privatizzato il sistema del *welfare* e in particolare il Sistema sanitario nazionale; lo abbiamo fatto rimanere accessibile a tutti e dobbiamo continuare a farlo.

è di 113 miliardi, quindi ci sono due miliardi in più rispetto a quello del 2015. È ovvio che facciamo i conti rispetto alla situazione economica, quindi diventa un dovere da parte di tutti noi fare in modo di eliminare gli sprechi, rendere efficace ed efficiente il sistema anche facendo azioni innovative, cioè entrando nel merito della produttività del sistema (in questo caso mi riferisco al senatore D'Anna), tant'è vero che nel piano di rientro che noi abbiamo inserito nella legge di stabilità non

le risorse non vanno più via, rimangono all'interno del comparto, con delle priorità: quest'anno sono stati i LEA e il farmaco per l'epatite C; nei prossimi anni lo saranno il personale sanitario, l'innovazione e la ricerca e l'accesso ai farmaci. Sulla farmaceutica ospedaliera (non su

cioè al fatto che avremo nuovi farmaci che ci permettono di guarire rispetto a malattie che fino a ieri erano considerate totalmente incurabili, noi dobbiamo rivedere e rimodulare i modelli di accesso, e anche di spesa e di gestione. Su questo stiamo lavorando in un tavolo insieme alle Regioni

la senatrice Taverna. Per quanto riguarda gli *screening* noi abbiamo avuto e abbiamo a disposizione 5 milioni di euro per il 2014 e 10 milioni di euro per il 2015, motivo per il quale continuiamo ad applicare il decreto ministeriale che abbiamo previsto per non perdere Abbiamo espresso parere favorevole alla proposta della senatrice Taverna; quando avrà terminato l'*iter*, noi la assorbiremo nel sistema, in modo tale da non perdere queste risorse e di poter ampliare gli *screening*, che fra l'altro fanno parte dei nostri obiettivi, non solo a livello

cuore e rispetto alla quale da tempo aspetto una risposta è cosa sta facendo il Ministero della salute per garantire la sicurezza dei sistemi informatici in chiave antiterrorismo e quanto siete impegnati sulla *cybersecurity,* visto che c'è un tavolo specifico che ne se ne sta occupando. Da tempo non riesco a ricevere risposte ma lei prossimamente avrà la bontà di darmele. abbiamo il problema della personalizzazione dei presidi, soprattutto per le persone che stanno a domicilio. Più che avere una risposta sull'enunciazione di principio, su cui sappiamo di essere tutti con l'accordo,

nonostante il mio intervento, anche accorato sotto il profilo antropologico, oltre che biomedico. Mi astengo quindi dal fare una qualsiasi riflessione sullo stato di soddisfazione o meno della risposta, nella certezza che lei

impostazione va incrementata, perché se lei pagasse a tariffe e a prestazioni, andrebbe a finanziare gli ospedali più accorsati e dove i medici sono preferiti dall'utenza. Le voglio dare due informazioni, più che manifestare il mio apprezzamento che, come lei sa, c'è sempre quando andiamo verso ragionevolezza e competizione (perché *cum petere* significa anche cercare insieme e la competizione è la più alta forma di collaborazione). La pubblicità del Servizio sanitario non deve essere confusa con il monopolio statale della gestione. Il servizio deve rimanere universale e gratuito, ma deve avere, al suo interno, elementi di competizione, perché il malato riceva il meglio di quello che il comparto della sanità pubblica, a gestione statale, e il comparto della sanità privata accreditata, a gestione privata, possono dare. *(Richiami del Presidente)*. Se lei non mette in competizione questi due sistemi e paga

ahimè - per tutte le altre stanno tenendo in piedi il Sistema sanitario nazionale. Sappiamo benissimo quali sono: sono le Regioni che hanno già fatto la *spending review* e che lavorano sempre per dare servizi nuovi ai propri cittadini.

sia culturalmente che deontologicamente in un protagonismo attivo su questa problematica, che credo potrà essere aggredita e quindi ben risolta solo con la collaborazione attiva dei professionisti.

Signora Ministra, vi è il timore che alcune malattie contagiose seguano i cittadini extracomunitari interessati dalle migrazioni verso l'Europa. Preoccupano, in particolare, i casi di poliomielite che potrebbero accompagnare i migranti in fuga da alcuni Paesi africani, asiatici e dalla Siria. La poliomielite, purtroppo, è una malattia virale acuta, altamente contagiosa e dalle gravi conseguenze, soprattutto di tipo neurologico irreversibile. Quei migranti provengono da Paesi in conflitto e nei quali, purtroppo, le scarse condizioni igieniche e il basso tasso di vaccinazione permettono la diffusione delle malattie contagiose. La vaccinazione rappresenta una delle misure di sanità pubblica più efficaci per la protezione della salute, sia individuale che collettiva (mi rifaccio all'intervento della collega che In tal senso le chiediamo, signora Ministra: se il sistema europeo di prevenzione contro la poliomielite e contro le altre malattie contagiose sia adeguato a garantire l'immunità della popolazione, ovvero se non sia opportuno rafforzare i sistemi di controllo e prevenzione; quali siano le misure che si stanno attuando e che si intende attuare per controllare i profughi extracomunitari, in particolare quelli siriani che entrano nell'Unione europea; se i bambini provenienti dai Paesi a rischio siano stati vaccinati contro il virus della poliomelite e sottoposti ad uno *screening* completo che escluda qualsiasi forma di incubazione del virus a lungo termine; quali iniziative intenda assumere al fine di estendere la vaccinazione obbligatoria alle persone non immunizzate in fascia di età avanzata e se non ritenga necessario intraprendere azioni conoscitive e campagne informative sull'argomento.

verso i medici e i pediatri, che devono ritornare al centro del sistema sanitario, verso la politica, che sempre più si è allontanata dal difendere gli interessi dei cittadini per rappresentare quelli dei grandi gruppi di potere, verso le case farmaceutiche, che trasformano la salute in profitto (e i farmaci per l'epatite C ne sono un esempio), verso il mondo scientifico, che ha abbandonato l'approccio della medicina basata sull'evidenza e si è lasciato contaminare da pubblicazioni con risultati spesso discordanti. I cittadini sono sconfortati nel vedere che il calendario riportato all'interno del Piano nazionale di vaccinazione è la copia fedele del Calendario per la vita sponsorizzato dalle industrie del farmaco e l'unica risposta che è stata data è una minaccia di querele. Gli studi preparatori per il Piano nazionale vaccini hanno visto come *sponsor* le stesse ditte che producevano vaccini ed il Piano è stato redatto, tra gli altri, dall'Istituto superiore di sanità e da quattro società scientifiche di cui non conosciamo neanche i documenti contabili, il Piano potenzia l'offerta di vaccini, spesso discutibile, rispetto ai cicli vaccinali di base, senza risolvere il nodo di come raggiungere le coperture necessarie a trasformare in salute questo potenziamento di offerta. I cittadini sono quindi sconcertati dai conflitti di interesse che si vedono a numerosi livelli. Per ridare fiducia a loro, le chiedo cosa ha fatto e cosa sta facendo il Governo. Le ricordo anche che, sull'argomento, il Movimento 5 Stelle ha presentato un'interrogazione, la

*(Misto-Idv)*. Signora Ministra, la campagna di vaccinazione intensiva contro il meningococco C, decisa a seguito dell'aumento dei casi registrati in Toscana rispetto agli anni precedenti, ha comportato la previsione di misure straordinarie di promozione della vaccinazione.

questa campagna si è tradotta in una vaccinazione a tappeto, sicuramente alimentata anche dall'allarme mediatico e sulla cui efficacia si potrebbe ragionare in maniera critica. Le mie domande sono molto semplici. Anzitutto, preso atto che i contagi sono avvenuti attraverso il contatto con un portatore sano, non sarebbe stato più utile avviare un'indagine epidemiologica che, attraverso l'utilizzo di tamponi faringei, fosse specificatamente finalizzata alla ricerca dei portatori sani? Per quali ragioni l'ipotesi di una indagine mirata non è stata presa in considerazione?

Cosa pensa il Ministero sulla introduzione da parte dell'Ordine dei medici di incentivi per i medici in proporzione alle vaccinazioni effettuate o, al contrario, di sanzioni per chi non vaccina? Questa, come ha evidenziato il collega Gaetti, è una cosa che mina molto

alla sensibilità chimica multipla e vorrei sapere quali siano le possibilità reali di inserire questa patologia, insieme alla fibromialgia, tra le malattie croniche invalidanti, cosa che molti cittadini ci stanno chiedendo, nonostante la difficoltà

non ribadisco le cose che hanno detto i colleghi sulle campagne vaccinali. Le dico però, per esperienza diretta, che c'è una *vulgata* che tende a ritenere inutili, se non dannosi, i vaccini, soprattutto perché causerebbero l'insorgenza dell'autismo. quindi opportuno che il Ministero facesse una controinformazione rispetto alla propalazione di queste notizie che sono del tutto fuori posto e fuori luogo. Le devo anche segnalare, però, il fatto che la gente non distingue più tra le vaccinazioni obbligatorie e quelle che giustamente, in questo caso con ridondanza,

mentre sono stati chiusi i centri privati accreditati che i requisiti li avevano. Signor Presidente, ricordiamo che, secondo la legge italiana, le vaccinazioni obbligatorie sono quattro, a cui si affiancano nove vaccini cosiddetti facoltativi o raccomandati. Il diritto alla prevenzione vaccinale oggi viene garantito, con splendidi risultati, in tutto il mondo occidentale, senza alcun obbligo di legge, ma con programmi di offerta attiva da parte dei servizi sanitari che prendono in carico il nuovo bambino arrivato. La Regione Veneto ha attualmente sospeso l'obbligo di vaccinazione sul suo territorio a fronte di un'offerta attiva di vaccinazioni che è tra le migliori in Italia e le prime in Europa, erogata attraverso una rete di servizi pubblici e una costante intesa con i pediatri di libera scelta. Va inoltre sottolineato che qualsiasi trattamento di tipo sanitario è, di norma, volontario e che l'Unione europea ha emanato una raccomandazione sul tema, proprio in riferimento ai vaccini. Si tratta di una novità che trova fondamento nel Piano nazionale vaccini 2005-2007, in cui è previsto un percorso per il superamento dell'obbligo vaccinale. Queste tredici vaccinazioni in molte Regioni vengono offerte gratuitamente attraverso i LEA. Il problema, però, è che la differenza che c'è tra Regione e Regione produce diseguaglianze di accesso e sprechi economici enormi. I quattro vaccini obbligatori hanno all'incirca una copertura

La domanda che rivolgiamo al Ministro è se, essendo a conoscenza della situazione, non intenda intervenire al fine di costituire un gruppo di lavoro formato dalle società scientifiche di pediatria e infettivologia allo scopo di promuovere linee guida basate sull'evidenza medica per garantire una maggiore assunzione di responsabilità del Servizio sanitario nazionale, condividendola però con i genitori che sono chiamati a rendersi partecipi nell'esigere il diritto del proprio figlio di non ammalarsi di malattie prevenibili col vaccino e non più, quindi, ad essere esecutori passivi di un obbligo imposto, nel qual caso si rischia un ulteriore calo delle vaccinazioni nei prossimi anni, come quello che

minuti anche se non è semplice, perché ognuna di queste domande meriterebbe una risposta estremamente approfondita. Sono debitrice dalla precedente interrogazione di una risposta - perlomeno lampo - per quanto riguarda la fibromialgia: siamo in attesa dei *cut-off*, e senza questo sarà difficile che riusciamo a inserirli nei LEA, nonostante dobbiamo dare assistenza alle persone che hanno questa sindrome. Per quanto riguarda riguarda la sindrome di sensibilità chimica multipla, tra l'altro una sindrome estremamente particolare, come sa l'interrogante, senatore Romano, si sono già espressi più volte sia il Consiglio superiore di sanità sia l'Istituto superiore di sanità. È veramente ancora complesso identificare la malattia in modo tale da poterla inserire all'interno dei LEA, però recepisco la domanda e anche la richiesta che viene dalle associazioni e quindi mi impegno a mandare una nuova richiesta di esame, per avere un aggiornamento dei dati scientifici attuali, al Consiglio superiore di sanità. Per quanto riguarda il tema dei vaccini che, come sapete, è uno dei temi che mi stanno più a cuore come Ministro, perché ritengo che le vaccinazioni siano l'ABC della sanità pubblica, ricordo a tutti una notissima vignetta dove ci sono due persone dell'epoca di Neanderthal, l'una vicino all'altra. Una dice: «Qualcosa proprio non va. La nostra aria è pulita, la nostra acqua è pura, tutti noi facciamo molto esercizio fisico, tutto quello che mangiamo è biologico, eppure nessuno di noi vive

politiche attive per vaccinazioni di massa, per mantenere l'effetto gregge nel nostro Paese. L'effetto gregge serve soprattutto per quei bambini che non possono essere vaccinati, o perché troppo piccoli o perché hanno patologie che non consentono loro di ricevere una vaccinazione, per permettere loro di scuola o in una comunità insieme agli altri bambini senza rischiare, a volte, purtroppo, la vita. Questa è la filosofia di fondo per cui noi dobbiamo continuare a fare informazione in favore dei vaccini e questa è la filosofia che ci ha portato al nuovo Piano nazionale vaccini, che - lo voglio evidenziare - è finanziato per circa 220

Come è stato detto dai colleghi senatori, molte vaccinazioni non sono obbligatorie, sono volontarie. È difficile per i cittadini tra vaccinazione obbligatoria e vaccinazione volontaria o facoltativa, ma questo fa parte di un approccio filosofico che ormai hanno avuto quasi tutti i Paesi occidentali dall'inizio degli anni Novanta. Il Piano nazionale prevenzione vaccinale vuole andare a incidere su questo, cioè sull'educazione e sulla formazione, non solo dei genitori dei bambini che devono essere vaccinati, ma anche degli operatori sanitari. È, quindi, assolutamente necessario un coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, dei neonatologi, dei medici di medicina generale, ossia di quelli che sono i soggetti attivi. Inoltre, partiranno campagne istituzionali, previste dal Piano nazionale prevenzione vaccinale, per la promozione della vaccinazione, ma anche per una corretta informazione delle famiglie rispetto ai possibili effetti avversi, che sono pochi, rarissimi, ma sui quali comunque, come per qualsiasi somministrazione di un farmaco, abbiamo una casistica. I genitori, quindi, devono essere preparati ad

indipendente ci permette anche di sfatare alcune situazioni o di avere una maggiore certezza su un processo che un grande Stato come il nostro non può far altro che favorire. A questo proposito, proprio il Centro nazionale per la inserito questo *topic* nell'ultimo bando che è stato finanziato su alcuni progetti. Inoltre, abbiamo dodici milioni di euro appositamente approvati nei bandi di AIFA, proprio per la ricerca indipendente, che prevedono di inserirsi in questo contesto. Infine, anche nel bando finalizzato alla ricerca del Ministero della sanità sono stati previsti fondi per la ricerca indipendente. Questo per dire che c'è una particolare sensibilità

purtroppo, abbiamo avuto casi precedenti negli ultimi anni. La malattia ha avuto un andamento di questo tipo negli anni e la Regione Toscana è intervenuta nell'area in cui in modo particolare si sono concentrati - anzi, si sono concentrati solo in quell'area - i casi di meningite con una vaccinazione di massa, secondo quelli che erano i criteri, cioè prima la fascia dei più piccoli, più piccoli, poi le fasce adolescenziali. Si è poi visto che mano a mano cresceva la possibilità di contrarre il batterio, finché si è arrivati alla decisione di fare una vaccinazione di massa. abbiamo seguito l'andamento di quello che avveniva in Toscana e sono stati decisi ed approntati degli studi particolari da effettuare, anche con il tampone alla faringe, sulle persone che venivano a sottoporsi alla

veramente notevole di cittadini, e stiamo seguendo l'andamento non solo della vaccinazione, ma anche degli studi che verranno approntati e che si stanno effettuando, anche su persone già vaccinate, per quanto riguarda quest'area. al tema della poliomielite e dei migranti, che mi è stato sottoposto. Abbiamo avuto sicuramente una certezza in questi anni: l'esperienza enorme che l'Italia ha acquisito sui flussi migratori. Probabilmente è una delle esperienze più forti a livello sanitario mondiale, Il primo punto è che i virus non girano sui barconi ma - ahimè - girano in prima classe, e abbiamo visto con ebola che è accaduto proprio questo. Il secondo punto è che l'Italia ha fatto un lavoro straordinario, motivo per il quale dovremmo vantarci a livello internazionale e rivendicare il lavoro

Abbiamo pertanto garantito una copertura non solo per i cittadini italiani, ma anche per quelli di tutta Europa, cioè dei Paesi in cui queste persone sono poi defluite. È a questo punto veramente importante che siano vaccinati i nostri cittadini e che le persone si sottopongano a vaccinazioni ed anche ai richiami di alcuni tipi tipi di vaccinazione dopo molti anni dall'ultimo vaccino, così come consigliato dal proprio medico. Un'ultima cosa a tale proposito è che abbiamo avuto a novembre un'importantissima riunione dell'OMS a Roma, voluta da noi, che ha previsto una Carta della salute dei migranti, che poi è stata portata ed approvata dalle Nazioni Unite, ovviamente approvata anche a livello europeo, per cui noi facciamo un fascicolo del migrante e lo seguiamo nei suoi spostamenti, avendo in questo modo non solo l'identificazione della persona, ma anche evidenza delle patologie o di eventuali vaccinazioni che la persona ha riscontrato o avuto nel nostro Paese o in altri *hub*. Ciò è estremamente importante per controllare il sistema salute e garantire le norme di igiene, dal punto di vista della trasmissione dei virus e di altro, su tutto il contesto europeo. Questa è stata un'iniziativa italiana, del Ministero della salute, che ha avuto riscontro a livello mondiale. Signor Ministro, mi ritengo soddisfatta. Sottolineo nuovamente l'importanza di seguire e continuare ad implementare

Agli argomenti che ho proposto, su come conquistare la fiducia dei cittadini, per motivi di tempo non si è risposto in maniera esaustiva. Comunque, credo che questo Governo non abbia la forza di andare a incidere sugli elementi che che vanno a influire sul conflitto di interessi, che abbiamo visto essere davvero molto forte e che sono altrettanto importanti per cambiare l'orientamento. Se non si incide su questo, credo che di strada ce ne sia da fare parecchia.

Signor Ministro, la ringrazio per quanto ci ha detto. Il professor Umberto Veronesi amava ricordare che il disastro della medicina italiana è avvenuto quando è entrata in ogni casa l'Enciclopedia medica, perché potenzialmente eravamo diventati 60 milioni di medici. Quello che gira su Internet è incredibile: non dovremmo neanche più prendere l'aspirina! La ringraziamo per la determinazione e per il lavoro che farà per queste generazioni e le prossime. Mi ritengo estremamente soddisfatta. Sono parzialmente soddisfatto. Devo evidenziare però due punti. Il primo, è quello che anche se noi mettiamo tutte le vaccinazioni obbligatorie - a parte che è un errore mettere quelle non obbligatorie insieme a quelle obbligatorie, soprattutto l'epatite a due mesi, che credo nessun bambino prenderà mai

cento; dovrebbero essere rivaccinati, però non sappiamo quanto dura la copertura perché non siamo dei soldatini, ma siamo uno diverso dall'altro.

Poi, senza ombra di dubbio, le vaccinazioni fatte in maniera logica sono utili, ma tenga presente che se diamo incentivi ai medici per vaccinare, resta difficile che un paziente non chieda: ma lei mi vaccina perché guadagna di più?

Sono soddisfatto della sua risposta o della sua determinazione sui vaccini. Il tempo non mi ha consentito di esaurire gli argomenti relativi in terza battuta, le dico che non solo i poliambulatori dove si fanno le vaccinazioni o le visite specialistiche non hanno il decreto di apertura e funzionamento, ma buona parte delle strutture pubbliche non trasmettono tramite SOGEI al MEF il riepilogo delle attività. Lei ha solo i dati delle strutture della sanità pubblica e privata accreditata. Visto e considerato che lei deve fare i conti con i signori del MEF,

e ci sono stati dieci morti. L'auspicio è che almeno sulle vaccinazioni non ci siano tagli alla finanza pubblica, altrimenti sarebbe veramente un disastro. UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signor Ministro, sono soddisfatto della puntuale risposta che lei ha dato al mio quesito. È proprio quello che auspicavo: una risposta rigorosa sotto il profilo scientifico, in una valutazione molto approfondita su un tema che interroga nell'ambito del quale le posizioni sono sicuramente controverse. Riaprire il tema all'attenzione del Consiglio superiore di sanità è quanto io le chiedevo e la ringrazio per l'attenzione che mi ha voluto riservare.